e i suoi Stati membri, dall'altra. L'Accordo è stato sottoscritto il 15 ottobre 2008 nell'ambito della più ampia disciplina delle relazioni economiche tra l'Unione europea e i 79 Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. Le trattative per l'individuazione di nuove modalità di cooperazione tra tali due gruppi di Paesi sono iniziate nel 1998 e hanno condotto nel 2000 alla sottoscrizione dell'Accordo di Cotonou nel Benin, il quale va rivisto ogni cinque anni. Nel 2005 la revisione è stata firmata a Lussemburgo, con limitate modifiche rispetto all'Accordo di Cotonou, affrontando le medesime materie della cooperazione politica, della partecipazione strutturata, della collaborazione per la lotta alla povertà, della creazione di relazioni economico-commerciali e del miglioramento della cooperazione finanziaria. L'Accordo di Cotonou precostituiva la base per la stipula di singoli accordi di partenariato economico con specifiche regioni geografiche dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per superare il preesistente sistema basato sulla previsione di tariffe speciali per determinati beni. L'unico Accordo di partenariato ad oggi portato a termine è quello oggetto della ratifica in esame, sottoscritto tra la Comunità europea e i 15 paesi del Cariforum, appartenenti alla regione caraibica.

Cuba - ancorché membro del *Forum* - non ha partecipato ai negoziati. Haiti, che in un primo momento preferì soprassedere a causa di specifiche difficoltà interne, ha firmato l'Accordo nel dicembre 2009. Tale strumento mira a ridurre progressivamente le barriere all'interscambio commerciale e a rafforzare la cooperazione tra questi Stati e l'Unione europea. la povertà e favorire la sicurezza alimentare, agevolando l'integrazione dei Paesi caraibici nell'economia mondiale ed incentivando gli investimenti. In conclusione, la Commissione propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

calendario, pur molto intenso, dei nostri lavori, per dire due parole relativamente a questo Accordo. Il problema principale che l'Unione europea ha nei confronti di quell'area

da un lato, il traffico di sostanze stupefacenti; dall'altro, uno strano atteggiamento di aderenza alle norme internazionali che alcuni di questi Stati, in particolare quelli anglofoni o comunque di colonizzazione britannica, hanno ogniqualvolta si ritiene che i principi di sovranità nazionale non possano essere sopraffatti - così alle volte hanno anche detto - dal diritto internazionale (mentre invece noi sappiamo che proprio sul diritto internazionale si può sperare di costruire un mondo che possa avere pace e sviluppo, come del resto articolato tra gli obiettivi di questo Accordo bilaterale). Per quanto riguarda il traffico delle sostanze stupefacenti, occorre quindi tenere ben presente che si va ad entrare in relazione commerciale molto più stretta con una serie di piccoli Stati, tra cui un territorio d'oltremare ancora che sono il luogo attraverso il quale passa buona parte della cocaina che poi arriva sui mercati europei. Occorre quindi, quando si entra in contatto con questi Paesi, che si facciano scelte non solo relativamente

materie prime, che nei secoli scorsi sono state tra l'altro anche al centro di una serie di guerre e che ancora oggi sono ampiamente utilizzate nei nostri mercati; altrettanto ricca

di permanenza di proibizione nei confronti del consumo e del commercio delle sostanze stupefacenti, dopo cinquant'anni dall'entrata in vigore della Convenzione del 1961, non ha portato un risultato positivo, e quindi forse, magari di concerto con questi Paesi, occorrerebbe avviare un dibattito circa un approccio diverso. Ricordiamo, ad esempio, che in Giamaica la cosiddetta *ganja* è una sostanza utilizzata anche in riti religiosi o comunque considerati sacri o di aiuto a una serie di pratiche spirituali: penso in particolare ai rastafariani, che la usano non per "sballo" o per intossicarsi ma per aiutare e sostenere la meditazione o anche l'avvicinamento spirituale a verità che magari noi non conosciamo, o non riconosciamo in quanto tali.

attenti ad utilizzare la pena capitale come pena esemplare per imporre una giustizia là dove, in effetti, la criminalità non dico che abbia posto serissimi problemi di sicurezza nazionale, ma sicuramente, in virtù del fatto che da lì passa buona parte della droga che arriva in Europa e magari anche negli Stati Uniti, è presente. La preoccupazione, che è raccolta nei due impegni che si chiedono al Governo, da una parte vuole che l'Italia, assieme ai *partner* europei, che sono gli altri contraenti questo Trattato internazionale, avvii da subito - è stato detto che il processo negoziale di questo documento è durato oltre 12 anni una *démarche* politica e anche una serie di iniziative diplomatiche, perché non soltanto si passi, dove esiste, da una moratoria di fatto ad una moratoria *de iure* relativamente alla pene capitali, ma che in occasione di un prossimo voto dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla famosa risoluzione che l'Italia ha portato avanti, grazie alle iniziative, in particolare di «Nessuno tocchi Caino» e del Partito radicale nonviolento transnazionale e transpartito, da 17 anni,

delle Nazioni Unite quando si tornerà a votare sulla risoluzione. Quanto al secondo, l'impegno è a valutare l'opportunità se arrivare, qualora dovesse essere imposta la pena di morte (e continuano, purtroppo, ad essere emesse delle condanne), ma soprattutto

firmano Trattati con dei Paesi la cui reputazione dal punto di vista del rispetto dello Stato di diritto, delle riforme democratiche, dei cosiddetti diritti umani è dubbia. Nessuno si frappone al rapporto diplomatico, politico, economico e commerciale necessario con tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite: molti dei presenti in quest'Aula hanno addirittura votato a favore della ratifica del Trattato con la Libia; oggi abbiamo mandato le nostre armi contro la stessa persona con la quale due anni e mezzo fa si andava a braccetto, si scomodavano le Frecce tricolori e si facevano marciare in divisa d'onore anche i nostri Carabinieri. Occorre quindi dare un segnale chiaro nel caso in cui si dovesse derogare al rispetto dei principi come codificati dai Trattati internazionali in materia di diritti umani. Coloro i quali buona parte degli ultimi cinquant'anni li hanno spesi per promuovere quegli stessi principi a livello internazionale devono assumersi la responsabilità di prendere in considerazione la possibilità di sospensione di un Trattato con Paesi che invece non rispettano i principi che universalmente

e in qualche modo sono più facilmente guadagnabili alla causa dell'avanzamento o del progresso del diritto internazionale rispetto ad altri Paesi, come quelli verso i quali oggi tutti insieme, con un'alleanza più militare che politica, stiamo cercando di portare un'ulteriore stabilità basata su una minore tirannia.

Presidente, intervengo per chiedere di aggiungere la mia firma e quella del collega Marcenaro all'ordine del giorno

di cooperazione dell'Unione europea e - quindi - nei finanziamenti dell'Unione europea verso questi Paesi. Voglio ricordare ancora a tutti che si tratta, sostanzialmente, di un Accordo

L'azione non può essere bilaterale - stiamo parlando di un Accordo multilaterale - e, quindi, ci impegniamo subito a promuovere in sede comunitaria le iniziative per quanto riguarda Paesi che dovessero eventualmente riprendere la condanna alla pena di morte. Se il senatore Perduca accetta la riformulazione proposta, il Governo esprime parere favorevole sull'ordine del giorno.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti: - che, in relazione alle risorse da versare all'Unione europea, gli articoli 13, 14 e 15 dell'Accordo non incidano sull'entità complessiva dell'onere, ma solo sulla sua composizione interna, senza impatti aggiuntivi sulla finanza pubblica; - che l'istituzione ed il funzionamento dei centri di informazione di cui all'articolo 86 dell'Accordo avvenga ad invarianza di oneri per la finanza pubblica; che sia esclusa l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Staio, qualora il Governo italiano - nel ruolo di parte attrice di una controversia connessa all'interpretazione ed attuazione dell'Accordo - chieda la costituzione di un collegio arbitrale, ai sensi dell'articolo 206 dell'Accordo medesimo».

che l'Italia dei Valori vigilerà sugli atti posti in essere a seguito della ratifica di detto Accordo. Per questi motivi, annuncio il voto favorevole, seppur condizionato, del Gruppo Italia dei Valori.

c'è un risveglio improvviso di tutti i Paesi tradizionalmente in via di sviluppo o sottosviluppati che si trovano al di là dell'Oceano. Alcuni di essi si sono sviluppati con una forza ed una velocità che non sospettavamo,

che l'Unione europea e altre organizzazioni internazionali cercano di canalizzare con degli accordi come quello di cui stiamo discutendo adesso, non è possibile continuare con interventi economici più più o meno in stile elemosina per tacitare questo o quel problema, che normalmente significa povertà per quei Paesi,

Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico, con due brevissime considerazioni. La prima riguarda l'importanza di questa, che non è una delle tante ratifiche bilaterali che che abitualmente il Parlamento approva, ma una ratifica - se così possiamo dire - particolarmente pregiata perché incrocia due assi portanti della politica estera del nostro Paese: mi riferisco alla grande politica estera, quella di lungo periodo, di lunga durata. Come i colleghi sanno, i pilastri fondamentali della nostra politica estera sono l'integrazione europea, la solidarietà transatlantica, il multilateralismo e quindi l'importanza delle istituzioni multilaterali, a cominciare dall'ONU, e poi l'apertura ai Paesi emergenti, innanzitutto al primo cerchio (i Paesi del Mediterraneo e i Paesi che confinano geograficamente con l'Italia) e, in una prospettiva più ampia,

e un atto di rapporto, di relazione, di solidarietà con i Paesi caraibici, quindi con una parte importante del mondo dei Paesi emergenti. Credo quindi sia un elemento estremamente importante

e constatiamo come sul versante della cooperazione allo sviluppo, mentre si va continuamente restringendo lo sforzo economico bilaterale dell'Italia, per ragioni di tagli di bilancio sui quali ci siamo intrattenuti in altre occasioni e su cui pertanto non torno (una politica, a nostro modo di vedere, assolutamente sbagliata e miope perché taglia una prospettiva invece di prevederne una di crescita e di sviluppo anche per il nostro Paese),

perché questo documento fu presentato all'inizio di aprile, nel vivo della crisi derivante dall'afflusso di migranti dalla Tunisia. Già allora, però, si proponeva con grande chiarezza la minaccia che il regime libico di Gheddafi ha espresso pubblicamente, rispetto a ciò che lo stesso Gheddafi ha definito l'utilizzo di migranti illegali come bombe umane nei confronti dell'Europa, dell'Italia e dei Paesi della riva Nord del Mediterraneo. I tre mesi circa trascorsi convalidano quella preoccupazione e i motivi sottesi alla presentazione di questo documento parlamentare rivolto al Governo perché assuma posizioni conseguenti. Alcuni passaggi, tuttavia, sono invecchiati a causa del trascorrere del tempo, e io ho appena depositato, signora Presidente, alcune modifiche che tengono conto di novità di cui il Parlamento, all'atto di deliberare, deve prendere atto. L'argomento di fondo di questo documento parlamentare, colleghi, è il seguente. Noi ci occupiamo della problematica della migrazione, e anche delle migrazioni di massa illegali, quasi sempre sull'onda degli eventi, del dramma e della emotività legata a questi eventi. Il punto che la mozione vuole mettere in rilievo, e che già una relazione trasmessa al Parlamento due anni fa dal Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, aveva evidenziato, è invece un altro, in particolare. Esiste, ormai, a livello internazionale un crimine organizzato, strutturato, asimmetrico rispetto alle modalità di reazione degli Stati, e anche delle stesse organizzazioni internazionali, che è la tratta degli esseri umani. Oggi, la tratta degli esseri umani è il secondo crimine più lucroso per le organizzazioni illecite, dopo il traffico di droga. Ed è destinato a crescere ulteriormente, e a condizionare in modo drammatico la vita di milioni di persone e la stessa coesione del nostro Paese, come dei Paesi europei e degli altri che vengono fatti destinazione e bersaglio di questo traffico. È chiaro che il traffico di persone ha finalità diverse, e motivazioni sessuali, di sfruttamento sessuale, minorile in particolare. In molti casi, il traffico di esseri utilizza la condizione di debolezza, di povertà, di indigenza e di soggezione in cui si trovano molte persone per farle utilizzare da organizzazioni e da reti criminali come manodopera per attività diverse, a sfondo di sfruttamento sessuale in molti casi, ma anche di accattonaggio di manovalanza sfruttata sino alla conduzione in schiavitù. È dunque un fenomeno gigantesco, che ha le sue regole, abnormi e perverse; e vorrei permettermi di segnalare ai colleghi senatori un paragone improprio, certamente, ma che può aiutarci a comprendere. può aiutarci a comprendere. Lo ha fatto anche la Commissione difesa del Senato, meritoriamente, con un documento che è stato sottoscritto pochi giorni fa dalla maggioranza e dalle opposizioni. Quando ci siamo occupati della pirateria in Somalia, ponemmo un problema fondamentale, oltre al fatto umanitario: di volta in volta si rapiscono persone, si sequestrano navi, si creano ricatti,

in pratica nella Somalia, priva di uno Stato, oggi si è costituito un vero e proprio contro-Stato, una potenza regionale che ha disponibilità finanziaria e che è passata dall'uso del kalashnikov a quello dei missili, dall'uso di barchini con fuoribordo all'uso di mezzi in grado di aggredire grandi petroliere, addirittura con sostanze repellenti per il controllo dei radar. Ormai è diventata un'industria, ed è molto difficile contrastarla. Il senso del nostro intervento, signor sottosegretario Mantica, proposto al Governo e all'Europa e alla comunità internazionale per un'azione molto più incisiva contro il traffico di esseri umani e i *network* criminali che lo gestiscono e lo organizzano, è volto ad intervenire all'origine, alla fonte di ciò che noi ci ritroviamo in molti casi a Lampedusa. Si tratta di meccanismi, di fenomeni complessi, esigenze ovviamente il ragionamento che sottosta a questo documento parlamentare, Presidente, è che occorre una forte collaborazione internazionale per colpire queste reti criminali che nel frattempo stanno incamerando enormi risorse, centinaia di migliaia di euro freschi attraverso i quali si rafforzano, migliorano i loro apparati logistici, la loro capacità di corruzione nei confronti degli apparati dei Paesi di transito o di quelli di imbarco dei migranti, e dunque diventano, nell'intero continente africano - ma è un meccanismo molto grande che ovviamente si realizza in tanti Paesi asiatici - un'autentica multinazionale del crimine, o meglio dei noduli di un tumore che diventa rapidamente metastasi perché si diffonde a livello globale. Il succo di questa mozione risiede nel punto 6) che chiede sostanzialmente al Governo, sul tema dei crimini contro l'umanità e dei compiti della Corte penale internazionale, di aprire finalmente

dobbiamo a maggior ragione intervenire con la cooperazione internazionale nei confronti dei trafficanti, che stanno diventando via via una potenza asimmetrica nella realtà, in particolare africana, che è quella che riguarda tutti noi. Siamo consapevoli che la Libia aveva sottoscritto un accordo con l'Italia, che aveva implicazioni anche scomode perché portava alla detenzione, in condizioni talvolta disumane, di migranti spesso eleggibili come richiedenti asilo, tema molto delicato e grave. Ma la Libia aveva creato con la collaborazione ufficiale col Governo italiano un meccanismo di filtro rispetto a questa migrazione e alla gestione illecita del traffico delle persone. Noi ci siamo accorti che questo è diventato un grave problema al momento dell'esplosione della crisi in Tunisia; poi gli accordi che il Governo ha stipulato con il nuovo Governo tunisino hanno permesso di tamponare nuovamente questa situazione.

Ciò configura un crimine, tanto più nel momento in cui centinaia di queste persone, a causa dell'intento criminale del regime di Gheddafi, sono morte nel Mar Mediterraneo. di quanto detto, la mozione n. 406, dopo una parte di analisi e di descrizione della problematica, impegna il Governo: a mettere in campo nuove iniziative dell'ONU per contrastare le minacce alla sicurezza internazionale, visti il ruolo e l'attività delle reti criminali transnazionali nella gestione di traffici di esseri umani verso l'Europa, con la collaborazione delle Forze di polizia, dell'*intelligence* e della cooperazione internazionale; a dare all'Italia una funzione di *leadership* in questo settore; a proseguire da parte del Governo italiano nell'azione diplomatica nella collaborazione bilaterale con i Governi dei Paesi di origine e di transito; a collaborare con l'Unione europea, l'Alto commissariato dell'ONU per i rifugiati e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni; a rafforzare il pattugliamento navale congiunto europeo anche attraverso l'agenzia FRONTEX, in raccordo con i Paesi terzi direttamente interessati; interessati; a valutare la possibilità di attivare, anche attraverso il Consiglio di sicurezza dell'ONU, i necessari meccanismi previsti dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale di demandare alla Corte situazioni nei Paesi di origine e di transito dei flussi migratori in cui si possano configurare crimini contro l'umanità a carico dei responsabili di traffico degli esseri umani. Si tratta di un passaggio giuridicamente, politicamente istituzionalmente importante. Infine, sul piano nazionale, la mozione chiede di affrontare in modo certo e rigoroso dal punto di vista umanitario la ricognizione dell'identità e dello *status* dei migranti, garantendo priorità e tutela ai richiedenti asilo politico e ai profughi di guerra; a implementare la *task force* governativa per la gestione dell'emergenza; ad istituire urgentemente la funzione in Italia del *National rapporteur* sul fenomeno della tratta, come previsto della direttiva europea 2011/36/UE,

angolazione. Quante persone, uomini, donne e anche bambini, sono morte in questi anni nel tentativo di attraversare il Mediterraneo? L'UNHCR calcola che, solo dalla fine di marzo di quest'anno, siano 1.200 i morti nel Mediterraneo. Si stima che circa il 10 delle persone che tentano la traversata muoiano in mare. Allora, la prima domanda è cosa stiamo facendo, noi e l'Europa, per fermare questa vera e propria strage, che fa forse più vittime di quanti ne facciano i conflitti armati e i bombardamenti. È una strage che non possiamo far finta di ignorare, perché destinata a continuare: questi numeri sono destinati a ripetersi. Naturalmente, tutti abbiamo ringraziato i protagonisti italiani del soccorso in mare (Guardia costiera, Guardia di finanza e Carabinieri) e i comandanti e gli equipaggi che hanno prestato aiuto, ma la domanda è: questo basta ed è sufficiente, o è necessario che l'Italia prenda un'iniziativa urgente ed immediata per mettere all'ordine del giorno

forse ricorderete che il senatore Pisanu, illustrando un rapporto sull'immigrazione, ci disse qui, con un'espressione molto chiara, che l'unica alternativa all'immigrazione irregolare era ed è quella regolare.

le persone a mettersi nelle mani dei trafficanti. Certo che c'è un elemento coercitivo, ma tale mancanza di alternativa e la volontà di spostarsi sono più forti di qualsiasi minaccia, spingendo le persone a mettere in gioco anche la propria vita, pur di fare questa scelta. Se si vuole combattere la tratta dei mercanti di morte di morte è necessario intensificare e rafforzare le misure repressive, ma dovremmo imparare da una lunga storia che il proibizionismo è una risposta sbagliata a tale esigenza. C'è quindi la necessità di intervenire attraverso misure immediate, che l'Italia può prendere e sulle quali può farsi promotrice di un'iniziativa europea.

Il 7 aprile il ministro Maroni è venuto in Senato a parlare degli accordi conclusi il 30 marzo ed il 6 aprile con il sistema delle Regioni, delle Province e dei Comuni per una gestione solidale dei flussi, in particolare di quelli provenienti dall'Africa in seguito agli sconvolgimenti politici e alla crisi aperta in quella regione. Oggi approfittiamo di questa mozione per chiedere conto al Governo

il Ministro dell'interno ha ricevuto una lettera firmata da due sindaci, Giuseppe Castania, sindaco di Mineo, del PdL, e Francesco Pignataro, sindaco di Caltagirone, del PD. Di fronte a questa

I ritardi accumulati negli ultimi mesi fanno sì che le normative italiane ed internazionali sulla protezione dei minori in quelle condizioni non siano rispettate.

Come ha rilevato il senatore Livi Bacci negli scorsi giorni, si tratta di una palese ammissione del fallimento della politica del Governo degli ultimi anni,

leva ancora sulla paura: evidentemente, la lezione di Milano, dove la paura che avete cercato di sbandierare è risultata controproducente, non vi ha insegnato nulla nel corso delle ultime settimane. Avete deciso di mettere su questo provvedimento

Libia. Certo, sulle missioni sarà svolta una discussione specifica, e di ciascuna andrà valutata l'effettiva utilità, su cui poi andranno misurate le scelte. Ma noi sosterremo in punto di principio una linea che è esattamente l'opposto di questa che oggi viene dalla maggioranza. Chiederemo cioè che in ogni missione italiana, in ogni missione internazionale ci sia una quota di risorse che sia destinata non solo all'aiuto allo sviluppo ma ad un vero e proprio aiuto umanitario; chiederemo che le risorse per gestire civilmente i profughi che vengono dalla Libia siano strutturalmente previste come una parte essenziale di quelle previste per l'intervento in Libia. Dovrebbe essere chiaro che ogni euro speso in questa direzione, ogni euro speso per i diritti umani e per la democrazia è un euro speso anche per prevenire le guerre, per evitare che l'intervento umanitario si scopra solo situazione ha assunto i lineamenti del dramma e dell'emergenza e la via militare appare l'unica possibile. L'Italia potrebbe giocare un ruolo importante sullo scenario internazionale se scegliesse di costruire una *leadership* in questo campo, nel campo appunto della pratica e dell'esercizio umanitario. Il nostro timore è che la vostra politica abbia rischiato e rischi di compromettere anche questa possibilità.

eviterò di proposito di farne una parafrasi. Conto di provare a condurre un'arbitraria ma agile considerazione su due maestri che hanno potuto che hanno potuto insegnare all'Occidente un modo di guardare in controluce i suoi rapporti con il resto del mondo, e in particolare con il Terzo mondo. La prima figura di riferimento è stata riportata all'attualità da un convegno recentissimo (19 e 20 maggio) all'Università orientale di Napoli che, grazie al cielo, anche senza i soldi che le sono stati tolti, è riuscita a condurre una riflessione su Frantz Fanon e «I dannati della terra». Che effetto fa oggi rileggere «I dannati della terra», a cinquant'anni di distanza dalla sua uscita? François Maspero lo pubblicò nel 1961. Certo, cinquant'anni sono passati, ma il testo consente ancora di condurre una riflessione critica e autocritica sui rapporti tra Occidente e Terzo mondo. In questo autore, che ha avuto una vita sofferente e brevissima, c'è fortissimo il senso dell'affrancamento dall'Europa: è l'orgoglio della *négritude*, la valorizzazione della differenza. Dice: non abbiamo più motivo di temere l'Europa; smettiamo dunque di invidiarla. Bisogna provare a ricominciare una nuova vita basata su altri schemi culturali e su altri progetti. Non possiamo fare dell'Europa un'imitazione caricaturale e oscena. e oscena. «I dannati della terra» è un vero e proprio manifesto per la decolonizzazione, con le asprezze di quel periodo, con le sue durezze: Fanon collaborò anche alla lotta del Fronte di liberazione nazionale algerino. Una visione ostile alle potenze coloniali, e direi forse addirittura più severa nei confronti delle *élite* indigene che si adattavano ad un tipo di rapporto compromissorio con le potenze coloniali stesse e quelle in via di dismissione. Uno dei suoi libri è intitolato: «Pelle nera maschere bianche», quasi a sottolineare un processo di asservimento che le *elite* locali assumevano nei confronti del potere esterno. In questo autore non c'è un linguaggio politicista e vi è anche un rifiuto degli schemi economicisti del suo recente passato e presente: adotta piuttosto un linguaggio esistenzialista, dialettico, umanistico. Non è tenero nemmeno nei confronti dei Movimenti di liberazione, che hanno vinto ma hanno anche perso, perché nel momento in cui si sono adattati ad una tattica di breve periodo hanno rinunciato anche a continuare a rappresentare le funzioni che avevano messo in primo piano. La seconda figura - è un solco diverso, ma in senso complessivo può essere considerata insieme - è quella di Edward Said, un palestinese americanizzato, senza Patria, che ha vissuto - come dice lui - sempre nel posto sbagliato. Con il suo volume "Orientalismo" del 1978 - e che la cultura italiana provinciale ha tradotto soltanto nel 1991 - Said ha prodotto una sorta di monumento compatto, teso alla definizione del modello culturale che l'Occidente ha imposto sulla categoria dell'orientalismo e ha demolito un punto fondamentale cui hanno collaborato anche tanti altri: la cultura come individuazione di un campo autonomo dalle logiche del potere e dalle lotte politiche dentro l'arena sociale. Cito qualche frase: «L'Europa non sarebbe potuta essere completamente la stessa senza la sua storia coloniale. L'idea antropologica di cultura è stata in gran parte prodotta dall'esperienza coloniale. Il colonialismo stesso era cultura, emersa dal laboratorio coloniale come scienza e strumento di governamentalità». una visione dell'orientalismo come pratica che unisce scrittori, autori, pittori musicisti, viaggiatori e naturalisti, come una sorta di enorme *corpus* di idee che l'Occidente ha creato per fotografare un Oriente, che secondo l'autore non esisteva o che perlomeno fungeva soltanto da punto di appoggio per questa sorta di visione costruita, artificiosa ma potentissima. Questo *corpus* di idee e di scritti ha costruito una storia dei rapporti tra Occidente e Oriente in cui il sapere e la cultura hanno funzionato come mezzo di dispotismo e controllo, come strumento di gerarchizzazione e assoggettamento, strumenti davvero fondamentali per l'incorporazione delle popolazioni e dei territori orientati nel progetto imperiale occidentale. Traggo dal testo un esempio: «La pratica universale di designare nella nostra mente uno spazio familiare nostro, in contrapposizione ad uno spazio esterno è un modo di operare distinzioni geografiche che può essere del tutto arbitrario. Uso qui il termine arbitrario perché una geografia immaginaria del tipo "nostra terra\terra barbarica" non necessita necessariamente che i barbari conoscano e accettino la distinzione; è sufficiente che noi costruiamo questa frontiera nelle nostre menti: nostre menti: loro diventano loro di conseguenza; la loro terra e la loro mentalità vengono considerate diverse dalle nostre. si configura così come una sorta di scienza trasversale dell'annessione e del dominio, una sorta di schema storico-ideologico che è diffuso in tutta la tradizione critica della cultura occidentale moderna, cui tutti hanno collaborato». Secondo l'autore, è una tradizione malata, costitutiva della stessa identità occidentale, sintomo di una sua malattia più profonda: la sua violenza ontologica costitutiva, che corrode alla base le sue pretese più nobili.

«Ricondurre una regione dalla presente barbarie alla precedente classica grandezza, insegnare per il suo stesso bene all'Oriente i metodi dell'Occidente progredito, subordinare e mettere in secondo piano la forza militare per porre in risalto un grandioso progetto di conoscenza da acquisire nel quadro del proprio dominio politico in Oriente; teorizzare l'Oriente, dargli forma, identità, definizione, con il pieno riconoscimento del suo posto nella memoria storica e della sua importanza nella strategia imperiale, del suo naturale ruolo di appendice dell'Europa; conferire dignità al sapere acquisito tramite occupazione coloniale, considerandolo un contributo alla cultura moderna, quando i nativi non erano stati consultati, né trattati, altro che per istituire nuovi campi di specializzazione; creare nuove discipline, suddividere, dispiegare, schematizzare, incolonnare, classificare, registrare ogni cosa visibile e, se possibile, anche invisibile; da ogni dettaglio osservabile trarre una generalizzazione e da ogni generalizzazione una legge immutabile della natura, il temperamento, la mentalità, i costumi, i tratti costitutivi degli orientali. Sono questi i tratti della proiezione orientalista compiutamente realizzati nella descrizione dell'Egitto».

In questo contesto critico di visione controluce di un problema di grandi proporzioni che coinvolge centinaia di milioni di soggetti, occorre fare da parte nostra uno sforzo di interpretazione sui fondamenti culturali di coloro che si muovono: occorre non solo registrare le quantità, le statistiche, i milioni di persone che si riversano tra di noi

Occorre fare poi una riflessione sulle migrazioni più recenti e anche sulle ultime rivolte popolari. Penso che in Europa siamo tentati di attribuire a questi movimenti una sorta di

Siamo propri sicuri che i soggetti giovani, soprattutto quelli più giovani (che si muovono più degli altri, sia nelle rivolte che dentro i fenomeni migratori), abbiano semplicemente adottato dentro di sé

interpretare con saggezza la complessità enorme dei processi demografici. Faremmo un gravissimo errore ad interpretarlo in senso eurocentrico. Noi dovremo fare lo sforzo di leggere dentro queste lotte, dentro questi comportamenti, l'autonomia e l'indipendenza dell'altro, interrogarci; e quando non sappiamo capire, non pensare che non c'è niente da capire, ma porsi il problema, anche se non possiamo dare subito una risposta. La saggezza dell'interpretazione politica delle cose sta soprattutto nel non dare per scontato che la risposta è quella che già vive dentro le nostre menti: le nostre menti hanno dentro di sé dei testi già scritti in caratteri già preparati; siamo tutti abituati ad una sorta sorta di ipertesto mentale che ci portiamo dentro. Dobbiamo fare lo sforzo di leggere questi fenomeni uscendo fuori da questo ipertesto, e farlo per davvero. Solo così, probabilmente, possiamo riuscire ad avere un atteggiamento più giusto.

Grazie,

sull'isola di Lampedusa. Fatta salva la solidarietà agli abitanti di quell'isola e a tutti i soccorritori, vale la pena aggiungere poche, davvero poche, considerazioni, perché sono state dette cose importanti. Come è noto, tutti i dati degli indicatori relativi confermano che il fenomeno migratorio non è né transitorio, né un incidente. La crescita delle presenze in Italia di cittadini non italiani, nonostante il sostanziale blocco di due anni dei flussi di ingresso e le politiche di allontanamento, dimostra che non c'è alternativa alla ricerca di un saggio equilibrio tra spinta migratoria dall'esterno e capacità di accoglienza. È evidente che occorre mettere in campo una politica che attenui la forza e l'invadenza di un'economia sommersa che resta il principale attrattore per l'immigrazione irregolare. La crisi in Nord Africa ha generato nel 2011, secondo i dati di «*Save the Children*», un flusso migratorio verso l'Italia e le sue coste molto intenso, con 39.560 arrivi, fino al 23 giugno, sulle isole di Lampedusa, Linosa e Lampione, contro i 70 dello stesso periodo dell'anno precedente.

2010», stilato dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifiugiati, parla di cifre contenute, in termini sia assoluti che relativi, rispetto ad altri Paesi dell'Unione europea. In Italia i rifugiati sono 56.397, gli apolidi 854, mentre i richiedenti asilo ammontano a 4.076 unità; si tratta di cifre molto basse rispetto ai principali Paesi nostri *partner* europei. C'è stato un momento nel quale l'UNHCR ha addirittura chiesto all'Italia di giustificarsi per come

sono i giovani morti e sepolti nelle acque del Mediterraneo. È stato detto che la democrazia sa mettersi anche nella pelle dei naufraghi in fondo al mare. Solo i sistemi democratici, colleghi e rappresentante del Governo, possono accogliere i rifugiati, i profughi e, perfino, gli irregolari, perfino, gli irregolari, perché sanno che non è la paura che fa innalzare il livello di difesa, bensì la sicurezza sociale, l'organizzazione del lavoro, la capacità di programmare. Nei 27 Paesi dell'Unione europea, il 4 per cento della popolazione, cioè circa 20 milioni, è extracomunitaria, mentre il totale di quella straniera è pari al 6,4 per cento, cioè 31 milioni di persone. Tornando all'Italia, i dati ISTAT dicono che la presenza degli immigrati è sempre più una costante che genera ricchezza per il nostro Paese: è un fenomeno con cui necessariamente si dovranno fare i conti, e quindi non più rinviabile, se vogliamo garantire una reale integrazione per i lavoratori immigrati e le loro famiglie. Tenuto conto dunque che che la presenza regolare di stranieri nel nostro Paese sarà sempre più stabile, lungi dal respingere, diventa invece urgente la tutela di questa grande risorsa, a cominciare dal riconoscimento del diritto di cittadinanza per gli oltre 900.000 minori immigrati, di cui 600.000 nati in Italia. Presidente, quando compiono 18 anni, non esistono più, diventano irregolari anche loro. Almeno sull'infanzia questo Parlamento, in questo Paese, in questa Europa, dovrebbe avere in programma misure idonee, anche perché in questi giorni, intanto che parliamo degli immigrati, dei morti e delle guerre, ci è stato raccontato che abbiamo tanti giovani nostri emigranti di alta qualità in giro per il mondo, i nostri laureati: quasi 400.000 negli ultimi 10 anni. C'è sulla bilancia del dare e avere, dell'uscire e dell'entrare nel nostro Paese, un grande valore umano. Siccome è presente il sottosegretario Mantica, voglio concludere con una citazione che sembra

in una mozione con cui avevamo raccomandato al Governo di farsi parte diligente affinché, nelle sedi opportune, a cominciare dall'Europa, si desse il riconoscimento dell'avvenuta indipendenza del Sud Sudan. In questi giorni pare che anche in Somalia si muova qualche cosa di positivo. Mi pare che l'Italia, esattamente in quelle due parti dell'Africa, possa esercitare un protagonismo che faccia fiorire Presidente, lo scambio, soprattutto di giovani, rende i futuri cittadini dei nostri Paesi cittadini del mondo. Saranno loro che, riconoscendosi e capendosi, costruiranno democrazia e pace.

pari a 700 milioni di euro, mentre quelle della Comunità europea, che finora non ha rispettato i patti, ammontano a 20 milioni di euro.

l'ha detto anche il collega Rutelli - che dietro tutta questa situazione c'è un traffico di carne umana: ci sono le formazioni della criminalità organizzata che vogliono sfruttare la democrazia esistente nel nostro Paese.

personalmente ho fiducia nelle azioni del Governo - un programma serio per i respingimenti, sia per il bene di questi poveri disgraziati, che per il bene del nostro Paese,

le leggi che le mozioni - anche se chiaramente qui si parla dei flussi migratori e non di un dibattito a 360 gradi sulla politica mondiale - non si pongono un problema che sia uno sulla radice di tutto ciò.

emergenziali che, in deroga a tutta la normativa nazionale, europea e internazionale, consegnano a un commissario straordinario dei poteri che quasi non ha neanche il Presidente del Consiglio, dovendosi in qualche modo confrontare con i suoi colleghi del Consiglio dei ministri ed eventualmente con le Camere:

di conflitto, di carestia, di povertà, di persecuzione di qualsiasi tipo. Non ci si pone però nessuno dei problemi per i quali la gente più o meno liberamente decide di lasciare il proprio Paese di origine. Non ci si pone neanche l'altro problema, che

Oggi nell'Africa subsahariana ci sono circa 860 milioni di persone: si ritiene che nel 2050 saranno raddoppiate, 1,7 miliardi, cioè più del numero dei cinesi che vivono oggi in Cina. fare? Vogliamo forse creare un'altra fattispecie di diritto penale internazionale per tenere a casa queste persone, con la speranza di mettere in galera quelli che le trasportano nella parte del mondo ricco, che le ha tenute in povertà con il protezionismo, sistematica alleanza con i loro dittatori e la chiusura di qualsiasi attenzione ai diritti umani di qualunque tipo? Credo che se delle consonanze queste debbano essere ritrovate negli atteggiamenti umanitari e di carità umana che si recuperano nelle mozioni dell'Italia dei Valori e del Partito Democratico - non purtroppo in quella presentata dal

che sono riusciti poi a scappare e fortunatamente, un po' per conto loro, un po' perché è stato dato loro, alla fine, un permesso di soggiorno temporaneo, hanno trovato una migliore sistemazione, senza creare nessun tipo di problema di ordine pubblico in Italia.

a Potenza, il centro, simile alla prigione di Guantanamo, per come ce la raccontano (più che per come in realtà sia), cioè di pessima qualità umana, è in fase di chiusura, a Trapani non è mai stato aperto. Per questa risposta emergenziale il Governo ha stanziato 10 milioni di euro. Cosa succederà di questi danari? Non vorrei che fossero impiegati per rafforzare il controllo delle nostre "frontiere colabrodo" perché andrebbero esclusivamente ad aumentare i relitti, oltre che le pene eventuali delle persone che stranamente non vengono mai catturate. Signora Presidente, desidero testimoniare la grande attenzione che il Gruppo PdL ha per questa problematica, certo non da oggi, e per sottolineare il difficile compito che ha il Governo italiano oggi di fronte all'Europa. Grazie, sono primo Vice Presidente della Commissione che si occupa di queste problematiche presso il Consiglio d'Europa: la Commissione immigrazione e rifugiati. Il tema è caldo, anzi rovente, non solo per la situazione di Lampedusa e dintorni ma per quanto sta accadendo in questi giorni in Turchia, dove si sta verificando un fenomeno simile a quello di Lampedusa e di altre parti dell'Italia. Va detto che il Consiglio d'Europa ha attivato diverse iniziative per cercare di monitorare, ma anche di coordinare, i Governi interessati a questo fenomeno al fine di dare una risposta corale dell'Europa, e non soltanto da parte dei Governi che sono al centro del problema. Nell'ultimo dibattito svoltosi solo mercoledì scorso a Strasburgo all'interno della Commissione che si occupa di emigrazione e rifugiati è emersa chiara la consapevolezza di tutti i Paesi partecipanti

con una delegazione del Consiglio d'Europa, su mia proposta, abbiamo visitato Lampedusa, arrivando non ultimi ma, comunque, assieme a molte altre iniziative di questo genere: cinque parlamentari, due giorni e mezzo di visita. Desidero ringraziare, a nome del Consiglio d'Europa, e della Commissione immigrazione

personale altamente qualificato che ha fornito ai commissari di cinque Paesi diversi e di cinque gruppi politici differenti risposte competenti, precise, direi anche accorate che hanno contributo a dare di Lampedusa e del problema un'immagine serena, ma anche grave. Abbiamo visitato, ovviamente, i due centri di accoglienza, quello principale e quello organizzato presso l'ex caserma LORAN con valutazioni inevitabilmente differenti per la qualità dell'offerta di accoglienza che viene prestata. Particolare attenzione è stata dedicata alla differenza di qualificazione dell'immigrazione, distinguendo tra l'immigrazione cosiddetta economica (prevalentemente quella dei tunisini) e l'immigrazione dei rifugiati che scappano da situazioni di pericolo e di guerre (quella dei subsahariani alloggiati prevalentemente nel centro-ex In tutti i casi la prima opinione dei commissari del Consiglio d'Europa è stata altamente positiva per lo sforzo, la buona volontà, per la decisione

limitatezza della possibilità di fronteggiare una nuova eventuale ondata di emergenza come quella di aprile, quando più di 6.000 profughi ed emigrati, tutti insieme, invasero l'isola. Questa è una raccomandazione che sicuramente sarà fatta nel mese di ottobre, quando discuteremo, in sede plenaria, Grazie,

proprio dalla Commissione immigrazione e rifugiati, in quanto considerata precaria, a fronte di evidenti difficoltà da parte delle amministrazioni comunali di farsi carico degli oneri relativi. Infine, una notevole attenzione viene riservata agli accordi bilaterali, di cui il Governo italiano è stato protagonista, prima assieme al Governo della Libia e poi a quello della Tunisia. Questi accordi sono stati considerati con molta soddisfazione da parte di tutti i Paesi europei come segnale di una possibilità emergente di evitare un accordo globale da parte del Consiglio d'Europa, o dell'Unione europea,

proprio per farne un esempio da trasferire ad altre situazioni. Per quanto concerne il dibattito odierno, il Gruppo del PdL è in linea (e io personalmente mi dichiaro in linea) con la mozione il senatore Rutelli, con qualche adeguamento e adattamento per quanto concerne particolari passaggi, di cui credo sia già stato trattato il contenuto con il primo firmatario. Comunque, ringraziamo tutti coloro che, sotto questo aspetto, contribuiscono a dare un'immagine concreta, serena e positiva. Vorrei concludere anche io rivolgendo un saluto e un ringraziamento al popolo di Lampedusa. Ogni contatto con quella gente è esemplare. In due giorni e mezzo di presenza, come delegazione dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, abbiamo avvicinato, anche privatamente, tutte le ONG che operano sull'isola, i rappresentanti

una sola parola di rifiuto, nell'impegno privato dei cittadini di Lampedusa, di farsi carico di un pesante fardello, che non è solo quello di accogliere in prima istanza direttamente gli immigrati e i profughi quando c'è l'emergenza, ma di vedere la propria economia, cominciando da quella turistica, gravemente compromessa da questa situazione di emergenza. Prima di partire, i rappresentanti degli albergatori ci hanno detto, fuori dai denti, che si è ormai alla vigilia della stagione estiva ma che non hanno una sola prenotazione: le poche pervenute durante l'inverno sono state tutte disdette di fronte ai nuovi flussi di sbarchi. Di questo, signor Sottosegretario, la prego di farsi carico (e la collega Maraventano l'ha già sollecitata, come vice sindaco dell'isola), perché è un aspetto assolutamente non secondario di questa emergenza: il futuro di Lampedusa e dei suoi cittadini.

esteri*. Signora Presidente, vorrei sottolineare che, in realtà, sono in corso tre dibattiti, che si intrecciano, perché sembra che l'argomento sia comune ma il taglio fornito all'aspetto politico delle discussioni dice chiaramente che le tre mozioni si intrecciano ma rispondono a logiche profondamente diverse. Cercherò di rispondere brevemente ad alcune osservazioni che sono state fatte nel corso della discussione generale, anche esprimendo l'opinione del Governo sulle mozioni che qui sono state presentate. Da parte dell'IdV è intervenuto il senatore Pardi, che ha sollevato un problema di carattere molto ampio, che certamente trascende i limiti del dibattito in quest'Aula, ma che comunque

dei risultati positivi nella lotta alla fame nel mondo e abbiamo avvicinato alcune decine di milioni di individui a un livello di sopravvivenza minimo,

che lo sviluppo economico e sociale è fino ad oggi ancora l'unico in grado di rispondere a questa necessità. Certamente Cina e India sono governate da sistemi fra loro profondamente diversi, inseguono anche obiettivi di grande sviluppo, ma seguendo due linee particolarmente diverse (voglio ricordare che la Cina rappresenta la più grande industria manifatturiera del mondo, mentre l'India punta sul terziario, su una evoluzione più di *software* rispetto all'*hardware* cinese), ma la risposta è lì. Questo nelle molte politiche che attuiamo nei Paesi del Terzo mondo, in via di sviluppo, nei Paesi che stiamo coinvolgendo nella globalizzaione ci dovrebbe da un lato preoccupare per gli aspetti di carattere culturale che comporta; dall'altro ci dovrebbe far prendere atto che, al di fuori dello sviluppo economico, non esistono al momento risposte. E anche gli aiuti che diamo

gli attenti analisti e chi segue queste cose proprio attraverso la demografia di quei Paesi avevano lanciato alcuni segnali di allarme. Quando andiamo incontro a Paesi, a realtà sociali nelle quali grosso modo la metà della popolazione - in qualche caso il 40, in altri il 38 o il 42 per cento - è fatta di persone che hanno meno di 30 anni o di 25, è ovvio che siamo di fronte a un mondo diverso dal nostro. Siamo di fronte a una realtà che non riusciamo nemmeno più a comprendere, anche perché evidentemente viviamo una realtà che purtroppo per noi presenta percentuali totalmente diverse: forse dovremmo parlare di *over* 60 da noi per raggiungere quelle percentuali. Allora, la demografia diventa un argomento di analisi e valutazione certamente, ma anche una politica. Occorre evidentemente, sia da parte sia da parte della comunità internazionale nei confronti dei Paesi terzi, sia all'interno della comunità internazionale nei Paesi cosiddetti sviluppati, capire che questo è un elemento di grande cambiamento che sta intervenendo nel mondo, di fronte al quale occorre mettere in moto dei meccanismi

E di fronte a una mancanza di speranza di vita, le reazioni sono diverse, anche quella di infilarsi su un barcone e di affrontare il mare per raggiungere l'Occidente perché comunque, senza una speranza di vita, una sola speranza, quella del barcone, diventa una possibilità.

l'occasione che mi è data per far sapere che il 9 luglio, giorno dell'indipendenza del Sud Sudan, sarò orgogliosamente a Jiuba a rappresentare il Governo italiano. Si tratta di una realtà che ci sfugge: un grande Paese come il Sudan va a dividersi.

il cui risultato non può neanche essere messo in discussione, visto che più del 98 per cento ha votato per l'indipendenza del Sud Sudan. Anche questo è un nuovo fenomeno politico che occorrerà osservare con grandissima attenzione: infatti, di Sud del Sudan nella realtà africana ce ne sono molti, e se questo meccanismo si mette in moto, al di là delle complicazioni di carattere generale riguardo a quel continente, se ne apre un'altra di carattere più strettamente politico, che certamente ci deve preoccupare. ci deve preoccupare - lo dico per inciso perché lo collego alla debolezza dell'Egitto - il fatto che il Sud Sudan sia sul Nilo, e il controllo delle acque del Nilo è in quell'area l'elemento principe. A noi mancano petrolio e gas, ma il problema dell'acqua nella realtà del continente africano è ancora un elemento discriminante per le linee politiche.

civile, che è stato dimensionato sull'ipotesi di 50.000 migranti in 60 giorni e che è gestito dalla cabina di regia nazionale presso la Presidenza del Consiglio).

invece rispondere con grande serenità che il Governo ritiene di aver mantenuto gli impegni e di aver avviato, secondo gli accordi che erano stati assunti anche in sede europea, un processo

tavolo costituito con la Protezione civile alla Presidenza del Consiglio. Lei ha invitato il Governo a calpestare il terreno dei centri di accoglienza: io, con un po' di demagogia, vorrei invitarla a

vita. Se qualcuno non lo sa, lasciare l'Eritrea, dove esiste la coscrizione militare obbligatoria fino a 40 anni, vuol dire passare dalla parte dei traditori. E se qualcuno ancora non lo sa, ricordare che la coscrizione obbligatoria vale anche per i sacerdoti e per le suore. E se qualcuno ancora non lo sa, vale inoltre per tutte le donne, per cui nessuna di loro può uscire a qualunque titolo dall'Eritrea.

al perché oggi, nel gruppo dei disperati che vediamo sui barconi, contiamo tanti eritrei, tanti somali e tanti sudanesi. Ci sono realtà che vanno affrontate politicamente in quella sede e di cui vorrei che questo Parlamento un giorno avesse la forza di discutere, per assumere atteggiamenti severi nei confronti di chi, anche in sede internazionale, ne sottovaluta le conseguenze umane e psicologiche. C'è una grande C'è una grande confusione, dovuta probabilmente anche ai tempi: penso alla mozione Rutelli, presentata ai primi di aprile, quando il fenomeno dell'immigrazione clandestina dalla Tunisia ancora prevaleva rispetto a quello dell'emigrazione di quelli che chiamo «i disperati della terra», cioè gli uomini, le donne e i bambini che fuggono dalla miseria, dalla fame e dalle dittature dell'Africa subsahariana.

dopo i nuovi accordi che sono stati siglati dal ministro Maroni, il fenomeno cosiddetto dell'emigrazione economica, o dell'emigrazione tunisina (pensiamo ai famosi 28.000 tunisini), possiamo definirlo come praticamente inesistente, oggi.

degli africani subsahariani, che cercavano di raggiungere il Nord Africa come punto di passaggio verso l'Europa. E vorrei aggiungere che molti di loro, decine di migliaia di loro, erano la parte

Noi dobbiamo comunque partire da una considerazione di fondo: chi mette su barconi che non sono nemmeno in grado di navigare (credo che molti di voi li abbiano visti) voi li abbiano visti) centinaia di persone, donne e bambini compresi, senza nemmeno lo scafista (perché bloccano i timoni in direzione Lampedusa) e li dotano solo di un satellitare

che lo strumento di per sé, soprattutto tenendo conto dei meccanismi previsti dallo Statuto di Roma, potesse essere un elemento retorico più che di carattere procedurale e operativo. Il Governo ha poi ritenuto di concordare con il testo originario della mozione Rutelli, perché comunque il richiamo alla valutazione della «possibilità di attivare,

una delle aree più calde, quelle delle quali dobbiamo preoccuparci, è la vasta area che va dal Mashrek fino al Maghreb. Quindi, se non ci sono obiezioni, ma non credo, aggiungerei anche questo

ringraziandola di questa ambizione, che forse è meglio presentarsi in sede internazionale per operare attivamente perché si formi questa polizia internazionale sul modello EUPOL, lasciando alla sede multilaterale di discutere chi debba avere la *leadership* dell'operazione.

dal sottosegretario Mantica, ma inviterei il Governo ad accettare a sua volta che il Parlamento gli richieda un ruolo di primo piano.

nonostante la brevità dei tempi, è stato piuttosto ampio. Ha ragione il Sottosegretario quando dice che è stato più di un dibattito, perché sono stati citati fatti e idee che in realtà non sono esattamente inerenti alle mozioni in oggetto: siamo arrivati a parlare delle missioni militari, della mancanza della cooperazione allo sviluppo, che dovrebbe essere la soluzione migliore al problema dei migranti, affrontando il problema direttamente sul loro territorio. Ciò vuol dire che il Senato ha una grande passione

pone l'accento non soltanto a livello nazionale sul discorso dell'accettazione, dell'integrazione e della soluzione dei problemi di coloro i quali hanno diritto a chiedere l'asilo nel nostro Paese in maniera celere ed efficace, ma vuole colpire giustamente il fenomeno della criminalità organizzata nordafricana, e anche mediorientale, che approfitta delle debolezze e dei problemi di queste persone per autofinanziarsi e finanziare quindi le attività criminali che esse svolgono, sia sul territorio di

oggetto, come le altre, una tematica di estrema rilevanza sociale che richiede un'attenta riflessione da parte di tutti noi. Come correttamente osservato durante l'illustrazione delle mozioni che abbiamo ascoltato e giudicato, la crisi politica e sociale che ha coinvolto sin dall'inizio dell'anno la quasi totalità dei Paesi africani che si affacciano sul Mediterraneo ha determinato ingenti flussi migratori verso il nostro Paese. Emerge immediatamente come la gestione dei flussi migratori di questi mesi si sia rilevata inidonea, soprattutto tenendo conto della gravità e dell'importanza della situazione, e comunque, a nostro avviso, non sufficiente. Si tratta, tra l'altro, di un fenomeno, spesso gestito e manovrato dalle reti criminali transnazionali, nell'impotenza oppure nella connivenza con la benevola tolleranza anche da parte dei funzionari dei Governi dei Paesi coinvolti dai flussi migratori, che necessita di interventi forti e veloci. Per rendersi conto dell'entità della situazione basta tenere conto che sul territorio dell'Unione europea vi sono più di 8 milioni di migranti irregolari o clandestini provenienti principalmente dall'Africa e dal Sud‑Est asiatico. Grazie, che «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalle legge»; testo unico stabilisce che in nessun caso può disporsi il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali,

tali ultime questioni noi chiediamo di migliorare sensibilmente le condizioni dei migranti sistemati nei centri di accoglienza, nei centri di identificazione e espulsione e nei centri di accoglienza dei richiedenti asilo, centri che oggi - lo dico per chi non li ha mai visti o per chi li ha visti

delle disposizioni, troppi sono stati i casi nei quali i migranti sono stati accompagnati coattamente dalla Capitaneria di porto, dalla Guardia costiera e dalla Guardia di finanza Guardia di finanza in Libia e in Tunisia, senza che sia stato compiuto alcun accertamento volto ad appurare se tra gli stranieri respinti ci fossero richiedenti asilo politico. è un dato preoccupante. Signor Presidente, cari colleghi, non dimentichiamo inoltre che le politiche poco rispettose dei diritti inviolabili dell'uomo sono state recentemente colpite altresì dall'intervento della Corte di giustizia europea che ha sancito che il reato di clandestinità può compromettere la realizzazione dell'obiettivo di instaurare una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio nel rispetto dei diritti fondamentali.

al fine di accogliere e meglio gestire l'arrivo di migranti sulle coste meridionali del Paese, monitorando e garantendo la sicurezza stessa dell'Italia da eventuali infiltrazioni terroristiche e malavitose al fine di ripristinare i fondi per la cooperazione e lo sviluppo. Non credo sia un aspetto che possa essere contrastante e contrastato da un pensiero del Governo: una mozione che tiene in conto il rispetto del cittadino e di quella persona che proviene da una situazione drammatica nel suo Paese.

fosse stato di insegnamento per il Governo, spesso troppo impegnato ad intervenire in una materia delicata come quella dell'immigrazione con politiche repressive e in palese contrasto con la Carta costituzionale e le normative comunitarie e internazionali a tutela dei diritti inviolabili dell'uomo.

Grazie, se un Paese come il nostro, lo ripeto al Governo, rispetta i diritti umani, dovrebbe anche rispettare le mozioni che sono state presentate sul punto del

La *ratio* delle mozioni oggi al nostro esame è quella di impegnare il Governo, sia a livello nazionale sia a livello comunitario, ad adottare le misure idonee a rendere migliore la gestione dei flussi migratori e le condizioni di vita dei migranti, nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo. Questo è ciò che vorrei fissare nella mente del Governo, nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo. Per questi motivi, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo, l'Italia dei Valori,

Signor Presidente, è già stato rappresentato da alcuni interventi di colleghi che mi hanno preceduto come il fenomeno della tratta di esseri umani rappresenti un grande rischio per l'Italia. Infatti, il nostro Paese continua ad essere meta di flussi di clandestini provenienti dall'Europa orientale, dall'Asia e, oggi, a causa degli eventi bellici che ci sono nel Nord Africa, soprattutto dalla costa Sud del Mediterraneo. Secondo un rapporto del COPASIR, in Libia, già precedentemente agli eventi bellici attuali, ogni clandestino determinava un giro d'affari oscillante tra i 3.500 e i 5.000 dollari, con coinvolgimento di operatori anche nei ranghi della polizia e nel Governo di quei Paesi. La Libia da tempo, e oggi più che mai, è interessata da consistenti flussi di clandestini, provenienti da Paesi limitrofi, che utilizzano il suo territorio quale area di transito per l'esodo con destinazione Europa, attraverso l'approdo iniziale sulle coste meridionali dell'Italia e, in particolare, della Sicilia. Il fenomeno è serio e grave ed esige di realizzare un costante monitoraggio della sua evoluzione al fine di predisporre con tempestività gli interventi più idonei ad un efficace contrasto. È indispensabile, infatti, dal nostro punto di vista, che il fenomeno, sempre più vasto e articolato, dell'immigrazione clandestina venga gestito ed affrontato anche sotto il profilo specifico della tratta degli esseri umani, in considerazione dei suoi effetti sulla sicurezza nazionale. Per queste ragioni non possiamo non condividere molti dei contenuti delle mozioni che oggi sono al nostro esame. Tuttavia, vorrei anche cogliere l'occasione per avanzare delle riflessioni a più ampio raggio. Ad oggi, in Libia permane una situazione di forte instabilità. Gheddafi, sintesi di equilibri di clan e tribali, sembra non volerne sentire di lasciare il potere e il suo Paese, oggi fortemente dilaniato.

A tre mesi dai primi sorvoli nella zona orientale della Libia, la NATO continua a bersagliare vari obiettivi lungo tutto il Paese. L'operazione militare, decisa e votata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha visto finora circa 5.000 missioni aeree da attacco condotte dai *jet* della NATO. Attualmente gli aerei dell'Alleanza colpiscono una cinquantina di obiettivi al giorno, la maggior parte a Tripoli, Misurata, Brega e nelle montagne di Nafusa. Per la prima volta un capo di Stato è stato deferito alla Corte penale internazionale, la quale pochi giorni fa ha emesso un mandato di cattura nei confronti del leader libico, del figlio primogenito e del capo dei servizi di *intelligence* di Tripoli. Persiste quindi una situazione grave di caos e incertezza. Ciò che emerge con tutta evidenza invece è come l'Europa si sia dimostrata sorda all'anelito di libertà proveniente dalla sponda Sud del mediterraneo e non abbia saputo prevedere con lungimiranza le richieste di cambiamento e di libertà. Ciò è imputabile alla lunga assenza di una politica per il Mediterraneo da parte dell'Unione europea. Risulta quanto mai necessario - quindi - recuperare lo spirito e gli obiettivi del processo di Barcellona e della politica europea di vicinato e sviluppare, contemporaneamente, un partenariato euromediterraneo in un rinnovato impegno di promozione di una politica di integrazione a tutti i livelli dei Paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo. Siamo di fronte ad un'occasione storica di corrispondere alle aspirazioni di tanti giovani, creando una casa comune euromediterranea, ove il rispetto delle tradizioni e delle culture possa essere il presupposto per creare qualcosa di più e di diverso in nome dello sviluppo civile, sociale ed economico, e dei principi democratici. È pura propaganda dire che interrompendo l'intervento NATO in Libia finiranno gli sbarchi sulle nostre coste. Gli sbarchi finiranno soltanto quando verrà ripristinata la pace e garantito un futuro ai giovani protagonisti del cambiamento. Come pure meramente propagandistico è il decreto approvato in Consiglio dei ministri: esso, tra l'altro, non fa che reiterare una proposta già avanzata da questo Esecutivo nel cosiddetto decreto sicurezza, che prevedeva già la proroga della permanenza nei CIE, rispetto alla quale lo stesso Governo fece a suo tempo retromarcia. Infatti, non è diffondendo la paura ma - al contrario - governando le emozioni e i fenomeni che si dimostra di essere classe di governo e classe dirigente responsabile. L'immigrazione è una ricchezza, se ben governata. Il 10 per cento del prodotto interno lordo viene, infatti, dagli stranieri. E' ora - però - che l'Italia appronti finalmente una seria politica sull'immigrazione. Non è possibile pensare di perpetrare soltanto una politica dei respingimenti. È bene ricordare che più del 70 per cento delle 31.200 domande d'asilo presentate nel 2008 in Italia provenivano da persone sbarcate sulle coste meridionali del nostro Paese, ma che, al contrario di quanto si pensa, solo il 10 per cento dei clandestini arriva via mare.

Su questo aspetto è necessaria un'operazione verità e politica. Questa potrebbe essere una grande occasione, che anche l'Europa deve saper cogliere, perché quello che sta succedendo nella sponda Sud del Mediterraneo investe anche il suo futuro e non soltanto il suo presente. Restringere la questione soltanto a quella migratoria sarebbe, quindi, riduttivo e miope. Di fronte alla latitanza dell'Unione europea, l'Italia è chiamata a fare la sua parte predisponendo le idonee risorse economiche e strumentali, nonché le necessarie previsioni giuridiche per affrontare l'emergenza flussi, onde garantire la sicurezza interna, contrastando l'immigrazione irregolare

i contenuti della mozione del senatore Rutelli, che invoca un pieno coinvolgimento dell'Europa e sollecita il Governo a procedere ad una rapida ricognizione dell'identità e dello *status* dei migranti già sbarcati in Italia, garantendo altresì priorità e tutela ai richiedenti asilo politico e ai profughi di guerra; a creare una *task force* governativa per la gestione dell'emergenza che metta al centro la fattispecie della tratta di esseri umani;

Grazie,

che vi sovrintendono, che stanno diventando una realtà imponente e decisiva, una minaccia che grava anche sul nostro Paese, e che tocca e colpisce la dignità di centinaia di migliaia di persone - perché, purtroppo, non abbiamo a che fare solo con migranti economici volontari,

Scrive il presidente Napolitano: «La comunità internazionale, e innanzitutto l'Unione europea, non possono restare inerti dinanzi al crimine che quasi quotidianamente si compie organizzando la partenza dalla Libia, su vecchie imbarcazioni ad alto rischio di naufragio, di folle disperate di uomini, donne, bambini.

di rappresaglia politica contro l'Italia e l'Europa. Ma è un crimine che si chiama "tratta" e "traffico" di esseri umani, ed è come tale sanzionato in Europa e perfino a livello mondiale con la Convenzione di Palermo delle Nazioni Unite nel 2000. Stroncare questo traffico, prevenire nuove, continue prevenire nuove, continue partenze per viaggi della morte (ben più che "viaggi della speranza") e aprirsi - regolandola - all'accoglienza: è questo il dovere delle nazioni civili e della comunità europea e internazionale,

del procuratore Ocampo di incriminare il presidente libico Gheddafi per crimini contro l'umanità, con riferimento al bombardamento di suoi concittadini

la gestione del traffico di esseri umani. Si tratta indiscutibilmente di una scelta innovativa dal punto di vista giuridico e di politica internazionale; è un fatto importante, che ovviamente non riguarda solo ciò che avviene in Libia, ma che fa

indispensabile riuscire ad intervenire con efficacia per prevenire e per collaborare con la comunità internazionale e con gli organismi esistenti, perché questi *network* criminali, che hanno in alcuni casi terminali

all'umana pietà non ci assolve, signor Presidente, se prima non siamo consapevoli che quei trafficanti bisogna contrastarli, perché stanno diventando un attore di prima grandezza sulla scena internazionale, stanno arricchendo e stanno influenzando i poteri istituzionali esistenti in molti Paesi del mondo. mondo. Non possiamo accorgerci della loro esistenza solo quando andiamo a contare i disgraziati che sono annegati nel Mediterraneo. Questo è l'oggetto principale della mozione sulla quale oggi il Senato si accinge a votare. Le altre mozioni producono e traducono sensibilità e focalizzano questioni diverse. Ci tenevo a chiarire che questa mozione risponde, direi quasi in modo pedissequo, all'appello che il Presidente della Repubblica ha riproposto più volte, e che il ministro Frattini ha rinnovato con grande efficacia, sottosegretario Mantica, quando a Napoli ha fatto appello alle nuove autorità libiche del Consiglio di transizione perché si facciano carico di questa problematica al momento di costituire un nuovo potere legittimo nella Libia *post* Gheddafi. Questi sono i temi davanti a noi e credo sia positivo che, seppure con un paio di mesi di ritardo rispetto all'attualità più urgente, il Senato li possa approvare oggi,

questo fenomeno

le armi». Dunque, al di là degli approcci un po' superficiali, banalizzati o demagogici che ho sentito echeggiare in quest'Aula, il problema del contrasto all'immigrazione clandestina via mare è un problema serio che va affrontato seriamente (l'onorevole Casini ci dice con le armi, sparando agli scafisti) e che, indubbiamente, questo Governo ha affrontato sin dall'inizio in maniera estremamente determinata, prova ne sia che l'attuale reato previsto dall'articolo 12 della legge Bossi‑Fini che colpisce gli scafisti, soprattutto i trafficanti di esseri umani, è stato modificato in senso ulteriormente repressivo da questo Parlamento, da questa maggioranza e da questo Governo. Oggi risulta quindi un reato particolarmente grave. Poi, se mi chiedete quante procure della Repubblica abbiano avviato indagini su questo tipo di reato, vi dico che i numeri sono davvero esigui, purtroppo. Noi possiamo lavorare, nel senso di dare tutti gli strumenti giuridici di contrasto, ma poi la magistratura è sovrana nel decidere se iniziare indagini su notizie di reato assolutamente irrilevanti, oppure su notizie di reato così importanti. condividiamo l'osservazione del sottosegretario Mantica, nel senso che questa maggioranza e questo Governo hanno già ben operato nella determinazione degli strumenti giuridici adeguati in materia di contrasto all'immigrazione clandestina per via marittima. Aggiungo che questo Governo, e il ministro Maroni in particolare, ha promosso forme avanzate di collaborazione internazionale. È stato ricordato l'Accordo con la Libia del 2009, che consentì di raggiungere risultati straordinari anche a vantaggio dell'intero territorio europeo. Si dice che ogni anno entrino in territorio europeo circa 400.000 stranieri vittime di traffico e di tratta. Ebbene, quell'accordo con la Libia riuscì

è poi il tema degli accordi bilaterali, che sono accordi sia di cooperazione di polizia di frontiera sia di riammissione nei territori di provenienza dei clandestini. L'accordo con la Tunisia, da ultimo stimolato, va proprio in questa direzione. Quindi, noi voteremo a favore della mozione n. 406 (testo 3) semplicemente perché è una mozione che auspica comportamenti da parte del Governo che il Governo ha già posto in essere in passato, che sta ponendo in essere e che porrà in essere per il futuro.

introducendo addirittura la categoria degli scafisti occasionali. Noi avevamo introdotto, nel pacchetto sicurezza del 2009, l'obbligo della custodia cautelare in carcere per gli scafisti. Quindi, c'era la possibilità dell'arresto obbligatorio in flagranza per gli scafisti, con la

sospetta di illegittimità costituzionale, perché gli scafisti non hanno tutti lo stesso ruolo e vi sono anche gli scafisti occasionali (sarebbe interessante capire da cosa sia determinata l'occasionalità dello scafista). Rimane il fatto che questa sentenza della Cassazione arriva dopo un'indagine delicata, che arrivò davanti al Tribunale della libertà di Roma, che nel 2010 confermò la custodia cautelare in carcere di quattro scafisti egiziani che avevano portato dei clandestini sulle spiagge di Latina. La

di piazza Cavour agiscono in maniera diametralmente opposta a quella che è una linea di indirizzo politico apparentemente condivisa da tutti gli schieramenti politici in questo Parlamento, allora diventa davvero difficile dare un contenuto serio alla lotta alla tratta degli esseri umani. apre una nuova finestra"). Colleghi, non lo dico per me, ma si manca di rispetto a quelli che intervengono in dichiarazione di voto. Vi è un'assoluta sproporzione tra rilievo del tema e serietà degli interventi e distrazione e brusìo continuo.

il grande tema dello sviluppo, o meglio della mancanza di sviluppo di un intero continente che è quello che cresce più rapidamente nel mondo. mondo. Di fronte a noi, a poche decine di miglia, si trovano le coste del Nord Africa, un'area - comunque si classifichi il Nord Africa - che conta tra i 150 ed i 200 milioni di abitanti, dove sono successe sollevazioni che non sono

erano tra un milione e mezzo e due milioni di immigrati provenienti dai Paesi vicini e dai Paesi dell'Africa saharianaa e sub-sahariana. Come tutti i grandi Paesi produttori di petrolio, la Libia vive e lavora perché c'è immigrazione. Vi è una altissima immigrazione come in tutta la penisola araba e questa immigrazione dovrà tornare una volta la situazione in Libia si sarà pacificata, non sappiamo se tra mesi o tra anni, ma dovrà tornare. E quindi, nuovamente, si ricreerà questo possibile serbatoio di immigrazione anche verso la nostra Europa.

persone che hanno valicato i confini della Libia, per metà verso la Tunisia, per un terzo verso l'Egitto e per il residuo verso i Paesi del Ciad, Niger, Sudan, Corno d'Africa e via dicendo. questa è la dimensione del problema: la Tunisia ha ricevuto quasi 600.000 transiti, in parte di tunisini che rientravano, in parte di cittadini degli altri Paesi africani; più di 20 volte il numero dei tunisini arrivati sul nostro suolo. E la Tunisia registra un sesto degli abitanti dell'Italia ed ha un prodotto lordo pari ad un cinquantesimo di quello dell'Italia. Dico questo per porre il problema nelle sue coordinate generali. Vengo ai problemi più concreti, quale quello del flusso attuale,

di queste ne voglio portare alla luce una: per esempio, l'atteggiamento del nostro Governo per quanto riguarda l'Accordo siglato a Napoli il 17 giugno scorso con il Consiglio nazionale di transizione libico.

che avrebbe firmato «un accordo sulla cooperazione per prevenire e contrastare i flussi di immigrati, inclusa la problematica dei rimpatri»,

Quale è la linea direttiva del Governo con riferimento alle migrazioni dei profughi? Qui c'è un grosso interrogativo, che naturalmente vorremmo fosse chiarito. Forse il ministro Frattini non si riferiva a tutti i 18.000 profughi dalla Libia ma a quelle poche decine di profughi che sono cittadini libici e che quindi forse, qualora non fossero minacciati di morte nel loro Paese, potrebbero anche essere considerati irregolari, e quindi rimpatriati. Vedete quale sproporzione c'è tra

"dobbiamo e possiamo considerare il cessate il fuoco come l'effettivo primo passo di una strategia politica di negoziato; un'immediata cessazione, o meglio una sospensione umanitaria,

comando italiano. In teoria, abbiamo la *leadership* formale per quanto riguarda il soccorso umanitario in Libia. Allora, qui domando perché non si spinga spinga la nostra autonomia di intervento a dare vita a EUFOR, che non può agire perché deve avere l'assenso delle Nazioni Unite, che però non è stato chiesto perché per agire dovrebbe intervenire con truppe di terra per proteggere i corridoi umanitari. Questo è il punto, Presidente: senza corridoi umanitari o senza presidi che permettano agli eventuali profughi di poter essere accolti e

fino al 2 giugno, hanno mietuto 1.615 vittime accertate nel Canale di Sicilia, senza parlare di quelle non accertate, che sono tante, come ci hanno spiegato i comandanti della Guardia costiera ieri, quando sono venuti in audizione nel Comitato Schengen.

per fare domanda d'asilo, bisogna arrivare sulle coste, o in un aeroporto o ad una frontiera del Paese nel quale si richiede l'asilo, ma se non ci si arriva, non si può richiedere asilo; si deve quindi tentare di arrivarci attraverso la navigazione:

ce ne toccherebbero 200.000, proporzionalmente al nostro peso economico e demografico, mentre ne abbiamo 56.000: la Germania invece ne ha 600.000 e la Francia 200.000. Concludo quindi confermando il voto positivo sulla mozione firmata dai senatori del PD ed anche un voto positivo di apprezzamento per alcuni

può avere la disponibilità del 95 per cento delle risorse mondiali. Viene anche in rilievo il problema della tutela della dignità umana: a distanza di molti anni dalla solenne dichiarazione dell'ONU del 1948, in cui si affermava che ogni individuo avesse diritto almeno al cibo, all'acqua, ai vestiti e ad una casa, quale effettività ha questa norma sul trattamento delle persone e sul rispetto della dignità e del valore umani? uomini dell'Occidente e noi italiani, che sul terreno della dignità abbiamo una cultura valoriale particolarmente accentuata dai principi cristiani che da 2.000 anni accompagnano la nostra storia, quale rilievo e quali politiche dobbiamo coltivare? Certo, c'è da domandarsi come possano attraversare mille chilometri nel deserto i profughi provenienti dalla Somalia, dall'Etiopia dal Centro dell'Africa; quanti bambini e quante donne riescano ad arrivare sulle coste del Nord Africa per poi essere trasportati dai trafficanti di morte e dai trafficanti di esseri umani in Europa, in Italia e, in

ragione che viene evidenziata in questa indagine. Sarebbe necessario valutare quale tipo di fuga da questi Paesi si profili: se si tratti semplicemente di persone che scappano dalla fame o se invece sia una fuga di cervelli, quindi questi Stati risultino ulteriormente impoveriti nelle loro risorse intellettuali, che invece potrebbero essere molto utili ai Paesi africani e nordafricani.

di alcuni funzionari o addirittura di alcune autorità di quei Paesi, ma sottolineo che essi richiedono un disegno organizzativo e criminale di vasta portata. La politica di cooperazione bilaterale e multilaterale risulta uno strumento ineludibile di cooperazione tra Stati, e probabilmente rappresenta per l'Italia

A mio giudizio, dovrebbe essere avviata una politica di cooperazione tra gli enti istituzionali della Repubblica. il nostro Paese è spinto verso un regime federale, in cui le Regioni hanno una potestà legislativa fondamentale, ad esempio in materia di assistenza e di servizi sociali.

non è un caso che l'articolo 117 della Costituzione abbia individuato nelle politiche di immigrazione, e in quelle di ordine e sicurezza pubblica le materie legislative che devono essere presentate al tavolo della cooperazione tra Stato, Regioni ed enti locali. Non mi convince, invece, la tesi sull'immigrazione illegale, posto che la maggior parte delle persone che vivono illegalmente nel nostro Paese non sono scappate attraverso le carrette del mare dal Mediterraneo.

di persone entrate nel nostro Paese tramite l'esenzione del regime del visto che alcuni anni fa l'Italia e gli Stati dell'Unione europea hanno adottato nei riguardi dei Paesi confinanti: dunque, tali persone sono entrate in Italia con il visto di ingresso per turismo o per studio e vi rimangono. Io ritengo che un precetto, quello di regolarizzare il permesso di soggiorno, sfornito di sanzione sia pura utopia:

si possa ragionare efficacemente sull'idea di ridare alla Corte penale internazionale e al diritto penale internazionale quella funzione che subito dopo la Seconda guerra mondiale, dopo i processi di Norimberga, si volle dare a quella struttura penalistica internazionale per contrastare e penalizzare comportamenti che andavano contro l'umanità, contro gli eccidi di massa, contro il nuovo fenomeno che noi oggi viviamo con le emigrazioni provenienti dai Paesi dell'Africa e del Nord Africa. Certo, il percorso del diritto penale sostanziale internazionale è stato travagliato, ma credo che noi italiani, che abbiamo visto qui a Roma sottoscrivere

pezzi di Stato che pensino che i diritti umani possano essere calpestati o vilipesi. Quindi, signor Presidente e onorevoli colleghi, portiamo il Popolo della Libertà a votare favorevolmente sulla mozione presentata dal senatore Rutelli in quanto siamo intimamente convinti che i valori della tutela dell'umanità, ma soprattutto della tutela della dignità umana, siano componente ed elemento essenziale dell'azione della maggioranza e del Governo, ma specialmente del rispetto di un popolo e del suo ordinamento, come il popolo italiano, che ha fatto di questi temi il centro essenziale della sua azione, e perché il nostro Paese possa dare un contributo fondamentale a questi temi,

per questo è stato creato lo scafista occasionale. La mozione n. 406 (testo 3) del senatore Rutelli, purtroppo, insiste nell'andare a colpire lo scafista occasionale o professionale senza porsi il problema dell'oggetto del trasporto. È per questo motivo che mi asterrò su tale mozione. Ultima questione: spero che il Governo abbia ben valutato il parere favorevole dato al paragrafo, seppur riformulato, relativamente alla Corte penale internazionale, perché non esiste quel crimine, nello Statuto di Roma. Quindi occorrerà, che alla prossima convenzione di revisione dello Statuto, l'Italia, ammesso e non concesso che possa avere sempre al Governo chi c'è oggi, dovrà proporre questa nuova fattispecie. Il problema dei flussi migratori sicuramente ha all'interno la lotta alla tratta degli esseri umani, ma non credo che questo debba essere il principale sforzo del nostro Governo per dare dignità umana a chi scappa, anche volontariamente e a proprie spese, da guerre e carestie. nuova finestra"). Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, permettetemi una breve cronistoria per inquadrare meglio il contenuto della nostra mozione. Più di trent'anni fa, con la legge n. 272 del 24 l'Italia ratificava la prima Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni, adottata all'Aja il 5 ottobre 1961. Il 19 ottobre 1996, circa 15 anni fa, nell'ambito della Conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato, veniva adottata la seconda Convenzione sulla «competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori», che aggiornava la precedente Convenzione del 1961 e che dava un contributo importante alla protezione dei minori a livello internazionale. A seguito della cosiddetta sentenza AETS della Corte di giustizia della Comunità europea in materia di competenza esterna, gli Stati membri dell'Unione europea non potevano più aderire individualmente alla Convenzione dell'Aja del 1996. Ne risultava una condivisione della competenza fra la Comunità e gli Stati membri, ma la Convenzione non prevede l'adesione della Comunità. Pertanto, il Consiglio europeo, con la decisione 2008/431/CE del 5 giugno 2008, autorizzava «in via eccezionale» quegli Stati membri che non avevano ancora provveduto ad aderire alla Convenzione «nell'interesse dell'Unione». In base alla citata decisione, per poter predisporre il deposito simultaneo degli strumenti di ratifica o di adesione, gli Stati membri interessati avrebbero dovuto scambiare informazioni

dopodiché il procedimento di ratifica avrebbe dovuto essere concluso simultaneamente, preferibilmente entro il 5 giugno 2010. La mozione oggi al nostro esame è stata da noi presentata il 3 novembre dell'anno scorso. Con essa non si chiedeva al Governo di procedere alla ratifica della Convenzione (pur essendo scaduto il termine da quasi cinque mesi), ma semplicemente impegnarlo a presentare il disegno di legge di ratifica. oggi, 29 giugno 2011, neppure questo minimo adempimento è stato posto in essere. Eppure l'importanza della Convenzione dell'Aja è universalmente riconosciuta tra i Paesi dell'Unione europea. Una volta ratificata, essa contribuirebbe a creare uno spazio giudiziario comune e permetterebbe di dare risposta ad un'infinità di situazioni problematiche, a tutt'oggi irrisolte, che vedono coinvolti migliaia di minori provenienti da situazioni familiari alquanto difficili. La Commissione europea considera questa Convenzione estremamente importante per la protezione dei diritti dei minori nelle situazioni di custodia di tipo internazionale e che coinvolgono più Stati. Come denunciamo nella nostra mozione, esiste il rischio che la Commissione europea possa attivare nei confronti dell'Italia la procedura contro la violazione dei Trattati, prevista dall'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dunque l'Italia sia costretta a presentarsi dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea e a pagare una probabile sanzione pecuniaria per il mancato rispetto del diritto comunitario. Non va dimenticato, tra l'altro, che l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, come modificato dall'articolo 1 del Trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2005, recita: «L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore». Come abbiamo specificato nella mozione, la Convenzione prevede provvedimenti di protezione del minore e dei suoi beni, escludendo l'adozione, gli obblighi alimentari e la sottrazione dei minori, già regolamentati da altre Convenzioni internazionali; definisce gli ambiti di applicazione stabilendo quale sia lo Stato competente e le autorità in esso esistenti che devono proteggere il minore nei singoli casi specifici, anche in riferimento alla localizzazione fisica dello stesso minore in un determinato momento, anche al fine di adottare provvedimenti di urgenza, determinare le leggi applicabili, garantire l'esecuzione delle misure di protezione del minore, cooperare con altri Stati coinvolti nel caso; prevede una procedura di consultazione da parte dell'autorità competente a disporre le «misure di protezione della persona e dei beni del minore»

ovvero quell'istituto giuridico di diritto islamico, presente nella maggior parte dei Paesi musulmani, attraverso il quale un giudice affida la protezione e la cura di un minore ad un altro soggetto (detto *kafil*) che non ne sia il proprio genitore naturale (nella maggior parte dei casi un parente), il quale curerà la crescita e l'istruzione del minore, istituto peraltro previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dei minori del 1989. Il Ministero dell'interno aveva posto inizialmente una riserva tecnica sulla *kafalah*, evidenziando la necessità di verificarne la compatibilità con l'ordinamento italiano e le esigenze di tutela dei minori. Tuttavia, il 22 dicembre 2010, nel corso dello svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata presso la Commissione esteri della Camera relativa all'argomento, il Governo, nella persona del sottosegretario Mantica, aveva dichiarato: «Ad ottobre, il Ministero dell'interno ha sciolto - limitatamente alla sola *kafalah* giudiziale (...) - la riserva in precedenza formulata. È stato così possibile convocare una nuova riunione dell'apposito tavolo di confronto interministeriale" presso il Ministero della giustizia. "A seguito di quell'incontro, il Viminale ha proposto una serie di affinamenti e di modifiche su alcuni punti del testo ancora in discussione. Quasi tutte le proposte sono state accolte dal Ministero della giustizia e si sta procedendo con il massimo impegno alla definizione di un testo finale condiviso. Considerata la comune volontà di tutte le amministrazioni coinvolte di condurre a termine positivamente il lavoro finora realizzato, è comunque prevedibile che (...) presumibilmente all'inizio del prossimo anno, sia possibile concludere le ultime e residuali verifiche tecniche e portare al Consiglio dei Ministri il disegno di legge di ratifica della Convenzione dell'Aja». Da quella data sono passati altri sei mesi. Crediamo dunque che i tempi siano davvero maturi

per la tutela dei minori: la convenzione de L'Aja del 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori;

importante adempimento; la mancata ratifica da parte dell'Italia di tale convenzione lascia dunque trasparire il debole interesse del Governo in carica per gli obiettivi specifici cui la convenzione è finalizzata, è finalizzata, di estrema importanza anche per il nostro Paese, e lascia ancora una volta senza risposte moltissimi bambini che aspettano di vedere riconosciuti all'estero, nel caso di trasferimento, i provvedimenti di protezione disposti dal proprio Paese di origine;

che integrano quelli relativi a materie già regolamentate, come l'adozione, gli obblighi alimentari, la sottrazione dei minori, e altre. Oggetto della Convenzione sono tutti i provvedimenti di protezione del minore e dei suoi beni, ad eccezione dell'adozione, degli obblighi alimentari e, come dicevo, della sottrazione dei minori. La Convenzione si applica in tutte le situazioni con elementi di internazionalità e ha i seguenti obiettivi specifici: determinare quale Stato è competente ad adottare le misure volte alla protezione della persona e dei beni del minore; determinare la competenza delle autorità del Paese in cui il minore si trova fisicamente per l'adozione di tutti i provvedimenti d'urgenza; determinare la legge applicabile dalle autorità competenti; determinare, in particolare, qual è la legge applicabile alla responsabilità genitoriale; garantire il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione del minore in tutti gli Stati contraenti; stabilire una cooperazione fra gli Stati coinvolti nell'emanazione e nel riconoscimento dei provvedimenti su minori. La principale novità rispetto alla Convenzione del 1961 consiste nella creazione di un'autorità centrale e nell'istituzione di una procedura di consultazione fra le autorità dei due Paesi di residenza attuale e di residenza futura del minore: ciò garantirà alle decisioni in materia minorile un riconoscimento il più possibile uniforme nei vari Stati, con il superamento del limite territoriale dello Stato in cui il provvedimento è stato emesso. La ratifica di tale importante Trattato consentirebbe al nostro Paese di dare finalmente una risposta a molteplici difficili situazioni che coinvolgono molti minori presenti nel Paese e che si trascinano da tempo senza alcuna soluzione; migliaia sono, infatti, i minori che vivono oggi, in Italia, in condizioni di difficoltà familiari: minori non accompagnati, bambini che provengono da Paesi colpiti da catastrofi naturali o conflitti, minori in *kafalah* (unico strumento di protezione e tutela dell'infanzia dei Paesi del Nord Africa) o in difficoltà familiare, che non sono ancora stati adottati. In particolare, il mancato riconoscimento dell'istituto della *kafalah* non consente ai minori abbandonati provenienti dal Nord Africa di essere accolti dalle aspiranti famiglie adottive in Italia; la Convenzione dell'Aja del 1996 aprirebbe, invece, la strada al riconoscimento delle misure di protezione che non hanno un corrispondente in Italia. La Convenzione, se applicata, avrà una portata storica perché permetterà di togliere da un limbo migliaia di minori in difficoltà familiare. Si tratta, infatti, dell'unico Trattato che si applica alla quasi totalità dei provvedimenti relativi ai minori in difficoltà e che è stato creato per contribuire a fondare uno spazio giudiziario comune. Questo è il punto fondamentale: si avrebbe, finalmente, uno spazio giudiziario comune. l'Italia è parte dell'UE, la quale ha interesse alla ratifica della richiamata convenzione in quanto si tratta di una convenzione di natura «mista», che per alcuni aspetti ricade sotto la competenza dei singoli Stati membri mentre per altri aspetti ricade nella competenza esterna esclusiva dell'UE nell'ambito dell'obiettivo della creazione di uno spazio giuridico comune all'interno dell'Unione (così la giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti tra i vari Stati dell'UE);

sottolineata, anche con petizioni che hanno raccolto migliaia di firme, l'importanza di tale Convenzione è stata richiamata con forza anche dalle 86 associazioni italiane attive per la difesa dei diritti dell'infanzia riunite nel gruppo di

In questi anni, a causa della mancata firma, l'Italia è già stata sollecitata dalla Commissione europea, che ora chiede ai Paesi dell'Unione europea di seguire il percorso fatto da molti Paesi, a partire da Spagna e Gran Bretagna.

al fine di attivare la procedura prevista dall'articolo 258 del medesimo Trattato contro la violazione dei Trattati. Esiste, quindi, il rischio che la Commissione europea attivi questa procedura contro l'Italia per la violazione dei Trattati, che prevede una fase giudiziale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee e che potrebbe anche comportare una sanzione pecuniaria per il mancato rispetto del diritto comunitario. Occorre anche ricordare ai membri del Governo che la mancata ratifica, inoltre, espone il nostro Paese al rischio di ulteriori sanzioni da parte dell'Unione europea e all'avvio di procedure che potrebbero comportare anche la condanna al pagamento di somme molto rilevanti. L'Italia non può più rinviare tale adempimento e deve procedere in tempi brevissimi alla ratifica della Convenzione in esame. Deve altresì approvare le norme necessarie all'attivazione delle procedure in essa previste, inclusa la nomina dell'autorità centrale, competente ai sensi della Convenzione stessa, strumento principe di diritto internazionale per la protezione dei diritti dell'infanzia a livello europeo e internazionale. insieme alle altre presentate, si vuole impegnare il Governo a presentare con la massima urgenza il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convezione dell'Aja del 1996

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ruberò solo pochi minuti per ricordare anche in questo ramo del Parlamento, com'è stato già fatto dal collega

quale ha partecipato anche il presidente Napolitano. Mi rendo conto che è ben poca cosa rispetto ai 150 anni dell'Unità d'Italia, ma si tratta comunque di un avvenimento storico che ha contribuito in maniera determinante determinante a cambiare l'assetto geopolitico del Centro Europa. Ovviamente, quella data ha significato anche l'inizio di un processo di disgregazione della ex Repubblica della Jugoslavia, con conflitti etnici, morti, genocidi, anche

per seguire poi con la Serbia, il Montenegro e gli altri Stati. In questa occasione, desidero ribadire gli ottimi rapporti esistenti tra l'Italia e e la Slovenia un po' in tutti i settori, rapporti che, come sappiamo, nel corso della storia, e soprattutto nel secolo scorso, non sono stati sempre facili: anzi, direi che sono stati improntati a

condivisi, che i due Paesi stanno affrontando insieme, in tutti i settori, da quello economico-commerciale a quello delle infrastrutture e della tutela delle rispettive minoranze. In questa occasione, desidero esprimere, a nome dell'Assemblea del Senato e dell'Associazione interparlamentare di Amicizia

mie felicitazioni per questo importante anniversario ed augurare a questo Paese, a questo giovane Stato di proseguire nel processo di modernizzazione modernizzazione e di innovazione che ha già dato ottimi risultati, visto che la Slovenia oggi è un Paese autorevole

è giusto sottolineare e apprezzare i rapporti positivi che oggi esistono tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia, che devono continuare e che, come lei stessa ha ricordato, sono stati testimoniati dalla presenza del Presidente della Repubblica alle cerimonie per l'anniversario. **Sulla Relazione

Se però si va a vedere in cosa consista la presentazione di tale Relazione al Parlamento, si scopre che si tratta della pubblicazione di due volumi, uno inviato alla Camera dei deputati, uno al Senato.

Contattando gli uffici della Presidenza del Consiglio si apprende che c'è un *link* al sito della Presidenza del Consiglio stessa, che però non sempre funziona. il tempo necessario un volume che spesso va oltre le 400 pagine, e tenuto presente che comunque, all'articolo 46 del Regolamento del Senato, si dice che le Commissioni

occorra prendere seriamente in considerazione questo problema. Annualmente siamo infatti di fronte all'impossibilità di confrontarci con il Governo circa i dati che vengono elaborati in questa Relazione. Lo si può fare solo un paio di mesi dopo, perché in effetti la mole di lavoro è tale che nei dettagli poi si scopre il diavolo. Si scopre infatti, per esempio, che i campioni sulla base dei quali vengono redatte le Relazioni è esiguo, per non dire ridicolo, e che sulla base di questa analisi antiscientifica si dice all'Italia che è diminuito il consumo delle droghe, chiaramente per rafforzare la necessità di indurire la legge cosiddetta Fini-Giovanardi e tutte le altre politiche di contorno, da ultima la gestione di oltre 13 siti *web* (neanche la Tunisia di Ben Ali aveva un sito *web* per un minimo aspetto della mera questione), che costano milioni, a dei nostri contribuenti. Fortunatamente, il sottosegretario Giovanardi risponde alle interrogazioni parlamentari e, quindi, abbiamo dati forniti dalla Presidenza del Consiglio. trovare un modo, e con la senatrice Poretti stiamo tentando di preparare un disegno di legge che ponga fine a questa prassi burocratica in merito a una questione molto importante. Occorre, infatti, ricordare che, purtroppo, 27.000 dei 67.000 detenuti nelle carceri italiane si trovano là in virtù della violazione della legge Fini-Giovanardi. Quando poi si va a vedere la qualità della violazione, scopre che si tratta dei cosiddetti pesci piccoli e che, all'interno di questo gruppo di pesci piccoli, la stragrande maggioranza, quasi il 65 per cento, non sono cittadini italiani. Il fenomeno è allora molto più complesso di quanto non si possa affrontare in una conferenza stampa di mezz'ora fatta da chi, chiaramente, non può che dare ragione a se stesso. Occorrerebbe forse che le Commissioni deputate, quindi Sanità e Giustizia, ma sicuramente anche l'Aula, affrontassero la questione nel dettaglio, magari con un minimo di tempo preventivo per potere studiare i dati, dal momento che poi ne conseguono tutta una serie di conferme e e ulteriori decisioni, che non sempre vanno nella direzione di gestire il fenomeno, ammesso e non concesso che l'obiettivo sia di gestirlo, piuttosto che rafforzare l'architettura proibizionista.

appropriata in sede di Conferenza dei Capigruppo, e non solo nelle Commissioni,il modo in cui su questo rapporto, con il tempo necessario, visto il tema certamente di rilievo che riveste, possa esservi un approfondimento non formale nelle Commissioni stesse e, eventualmente, in Aula. Su questo tema,